Signor Presidente, illustri colleghi, prima di esprimere il parere a nome del Governo, permettetemi di dare un contributo al dibattito avviato nella giornata di ieri. Il tema è la prevenzione ed il contrasto di fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione. Un tema - ha ragione il senatore Santini - sul quale non si può non essere d'accordo. Il problema non è dunque se, cosa o quando, ma come. La corruzione è un fenomeno radicato che - a nostro avviso - ha cambiato profondamente passando da una natura endemica, principalmente alimentata dalle costose strutture dei precedenti partiti-apparato, a fenomeno individuale a carattere plurimo, certamente assai diffuso, troppo diffuso, e purtroppo anche radicato, ma senza le caratteristiche di contiguità con il sistema politico che ha caratterizzato la cosiddetta Tangentopoli. Questo Governo è nelle migliori condizioni di impermeabilità alla corruzione per agire efficacemente, non perché il suo leader sia un uomo facoltoso, ma perché il suo leader è un uomo che gode di un amplissimo consenso popolare, più volte e recentemente riconfermato, che non ha davvero alcun bisogno di essere alimentato da forze diverse da quelle dei fatti e dei risultati. Il tema della corruzione è emerso in circostanze temporali pre-elettorali: non voglio dire per motivi pre-elettorali, ma certamente in circostanze pre-elettorali. La risposta del Governo è stata comunque pronta, specifica, articolata, ed è stata espressa dal disegno di legge approvato durante un Consiglio dei ministri straordinario dedicato a questo tema. I contenuti ne sono stati resi noti e sottoposti, nelle loro linee fondamentali, al giudizio della gente: un Piano nazionale anticorruzione, una Rete nazionale anticorruzione composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, nuovi obblighi per le pubbliche amministrazioni e per le stazioni appaltanti e misure sulla trasparenza che incidono su tre dei settori maggiormente a rischio corruzione: appalti, contributi, assunzioni. Poco tempo dopo, il corpo elettorale in elezioni amministrative, dunque particolarmente adatte a capire se vi è la conferma o il rigetto del consenso sulla gestione della cosa pubblica da parte di una classe politica, ha espresso un giudizio che mi pare chiaro e sul quale non è necessario tornare per decifrarne il segno. Sono la prima a dolermi del fatto che il disegno di legge non è ancora pronto in tutti i particolari per essere presentato in Parlamento. Si tratta di un'iniziativa interministeriale complessa e per molti aspetti innovativa che è in corso di definizione per taluni profili, specie concernenti la pubblica amministrazione. Se la corruzione d'altronde è il cancro del Paese, come ha recentemente titolato la stampa con una certa eco nazionale e come ancora ieri ha ripetuto il senatore D'Ambrosio, non si può non sapere che la cura per un cancro non sempre è semplice, né immediata, né purtroppo indolore. Se invece, come dicevano i senatori Benedetti Valentini e Gustavino, la corruzione è un'espressione patologica che si alimenta a partire da malcostume ed illegalità radicati - ed io sono in gran parte d'accordo - la conclusione non cambia: per un fenomeno con caratteristiche sistemiche serve una risposta di sistema, articolata su prevenzione ed informazione, non solo sull'aumento della repressione puramente edittale. Se il Governo avesse voluto fare un gesto solo simbolico avrebbe potuto limitarsi a questo; ma l'intenzione del Governo è sradicare il fenomeno, non tagliarne alcuni rami. Quelle stesse preoccupanti dimensioni del fenomeno che sono state citate nelle mozioni, e che evidenziano una situazione diffusa e radicata, testimoniano al contempo una situazione la cui responsabilità travalica di decadi la responsabilità di questo Governo: un Governo che è nondimeno convinto, e lo ha dimostrato, che debba essere messo in campo un impegno forte, un impegno deciso, un impegno concorde. Un impegno che coinvolga auspicabilmente tutte le componenti del Paese, senza distinzione, perché questa deve essere la battaglia di tutte le persone oneste. Rispetto a questo, gli atti di indirizzo su cui oggi il Senato è chiamato a votare sono, ad avviso del Governo, un'occasione perduta. Non per i contenuti: su parte dei concetti espressi nei testi che sono stati presentati vi può essere l'adesione del Governo. Diversi profili di indirizzo che risultano dalle mozioni si muovono lungo la stessa direzione verso cui si sta muovendo il Governo: penso, tra l'altro, alla necessità di sancire l'ineleggibilità per comportamenti accertati di corruzione, alla indispensabilità di un'efficace rete di informazione e di supporto all'azione sia preventiva che repressiva, al coinvolgimento del ruolo di tutte le componenti dell'amministrazione e in particolare degli enti locali. Tutti aspetti contenuti nelle mozioni. Ma dietro questi temi, non solo per come sono stati introdotti nel dibattito parlamentare dalle mozioni dell'opposizione, ma soprattutto per come sono stati sviluppati negli interventi, altri temi si sono ben diversamente manifestati. Lo ha detto il senatore Pardi, con una franchezza che apprezzo. «Non bisogna - ha detto - aver paura di essere reticenti: dietro questi atti di indirizzo, dietro questo dibattito parlamentare c'è chiaramente la figura del Presidente del Consiglio, l'azione di governo, le riforme che sta portando avanti, specie in tema di giustizia» C'è perfino - è stato evocato - il presidenzialismo. Lo dico chiaramente, signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori: non si può e non si deve fare della lotta alla corruzione un pretesto. È un tema troppo serio, è un tema troppo importante per farne terreno dell'ennesimo «no» politico globale e pregiudiziale. Deve essere soprattutto chiaro che la lotta alla corruzione non si fa con la guerra al garantismo. Perché se il punto è che il disegno di legge sul processo breve ostacola la lotta alla corruzione - e ricordo a me stessa

Ancora, se il punto è che il disegno di legge sulle intercettazioni ostacola la lotta alla corruzione, io dico che quel disegno di legge è un'ulteriore norma di civiltà giuridica, perfettibile quanto si vuole, fermo restando che non può proseguire in alcun modo lo scempio mediatico che si consuma con intollerabile frequenza e che alimenta un malcostume quotidiano in cui ci si abitua alla sistematica violazione del segreto istruttorio: un'abitudine alla illegalità che, come è stato detto, è anch'essa causa di malcostume. Ripeto, non si può fare e non si deve fare della lotta alla corruzione un pretesto. La lotta alla corruzione deve essere un impegno comune, e spiace che non si sia ricreato in quest'Aula quello spirito che ha consentito pochi mesi or sono una sia pur complessa convergenza sul tema delle riforme istituzionali. Queste sono le ragioni che motivano il parere favorevole sulle mozioni n. 263, presentata dal senatore Benedetti Valentini e da altri senatori, e n. 265, presentata dal senatore Mazzatorta e da altri senatori, ed il parere contrario (sebbene vi siano, come ho detto,

nn. 241, presentata dal senatore Belisario e da altri senatori, e 267, presentata dal senatore Rutelli e da altri senatori, e sull'ordine del giorno G1 presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri

come la meritano i presentatori delle mozioni in esame per avere richiamato l'attenzione del Parlamento su un tema che ha appassionato il Paese anche nelle ultime settimane, soprattutto nel periodo più a ridosso delle elezioni)

la discussione di merito sul disegno di legge che il Governo ha presentato e approvato in Consiglio dei ministri il 1° marzo recante misure e norme

sia l'osservatorio sulla corruzione e sugli atti illeciti contro la pubblica amministrazione, che verrà istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, nonché misure complessive sulla trasparenza, che completano quelle già adottate con il citato decreto legislativo n. 150,

Grazie, su una materia quale la corruzione che nasconde sotto questa unica denominazione fenomeni abbastanza diversi tra loro, sia per come si presentano e si configurano, sia anche per come si manifestano in alcune aree geografiche. È di tutta evidenza pertanto che questi spunti non andranno perduti;

Grazie, signor Presidente. che insieme agli amici del Partito Democratico abbiamo presentato proprio al fine di offrire un contributo propositivo. Voglio dire senza polemica che in questi giorni si discute, e parecchio, della riforma della giustizia e da parte di ampi settori della maggioranza

offerto, ritirando le proprie mozioni e convergendo in un ordine del giorno che sintetizza alcuni punti che peraltro sono stati espressamente indicati dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno nonché nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio come elementi qualificanti della lotta alla corruzione. Prendiamo pertanto atto con meraviglia

neanche nelle mozioni di maggioranza quali disposizioni di legge volete modificare, le norme che volete introdurre, le *Authority* che volete creare, ciò significa che c'è qualcosa che non funziona al vostro interno.

la vostra classe dirigente, anche in sede locale, orientandola verso modelli di comportamento conformi a principi di decenza amministrativa. Questo è lo scenario

Grazie, signor Presidente. Stavo dicendo che esiste una differenza di fondo sul piano delle motivazioni politiche, e anche culturali da un certo punto di vista, rispetto alle premesse della mozione dei colleghi dell'Italia dei Valori, sulla quale il mio Gruppo si asterrà, perché la chiave di lettura del fenomeno non può essere sempre e comunque ricondurre la lotta politica ad uno scontro da tenersi anche nelle aule giudiziarie, perché altrimenti questo Paese non uscirà mai dalla situazione di anormalità in cui si trova. Ci sono comunque alcune parti della mozione che noi condividiamo e che sono contenute anche nell'ordine del giorno che abbiamo presentato e nelle nostre mozioni; per questo,

non lo si è, ciò vuol dire che politicamente voi siete contrari, ad esempio, ad introdurre la confisca dei beni che siano frutto della corruzione.

Siete contrari, voi, ad estendere, ad esempio, ai più gravi reati di corruzione il sistema delle intercettazioni, così come previsto per i reati antimafia. Ci sono ben quindici punti in questo ordine del giorno, così come nelle altre mozioni,

ad una velina della Presidenza del Consiglio, ad un deliberato assolutamente privo di alcun contenuto, fatto il 1° marzo, più di un mese fa, le vostre sorti future sulla lotta alla corruzione. Credo che questo

credo sia, ad esempio, scandaloso che ancora oggi la Giunta per le elezioni del Senato non si sia occupata del rogo delle schede in Venezuela, perché questo fa parte di quei fenomeni corruttivi. Siccome peraltro la vicenda riguarda - come sembrerebbe da alcuni articoli di stampa - una collega del nostro Gruppo parlamentare, la senatrice Giai, di questo tema io investirò formalmente il Presidente del Senato. È infatti una vergogna e uno schifo che si brucino le schede elettorali da parte di organizzazioni criminali

l'intera classe dirigente eletta all'estero come un pugno di delinquenti per coprire quelli che sono realmente delinquenti, e lo sono in Italia, non all'estero. Questo non potrà più essere consentito a nessuno! Per queste ragioni, signor Presidente, noi voteremo contro le mozioni presentate dai colleghi di maggioranza, ci asterremo su quella di Italia dei Valori e voteremo a favore della mozione, che peraltro abbiamo sottoscritto, del senatore Rutelli; ovviamente voteremo a favore del nostro ordine del giorno, sottoscritto con i colleghi del Partito Democratico, forse responsabile ma non apprezzati dalla maggioranza.

colleghi, rappresentanti del Governo, leggevo questa mattina un quotidiano che nell'*incipit* scriveva così: «Dopo il roboante annuncio del primo marzo, dopo la solenne conferenza stampa dei ministri Alfano e Brunetta, dopo la presentazione ai giornalisti di questo disegno di legge governativo, o il disegno di legge anticorruzione si è corrotto oppure è stato corretto». Sta di fatto che al Parlamento questo disegno di legge non è ancora arrivato e anche le parole del sottosegretario Alberti Casellati sembrano più la prefazione ad un libro anticorruzione che l'annuncio di un provvedimento che la maggioranza vuol veramente adottare per la lotta alla corruzione. Il problema della corruzione (noi del Gruppo dell'Italia dei Valori abbiamo voluto con forza incardinare questa discussione in Parlamento)

Le cronache degli ultimi mesi, indipendentemente da quello che sarà l'accertamento sulle responsabilità che sono - come sappiamo - personali, hanno riproposto con tutta evidenza il tema della corruzione politica e del decadimento della vita pubblica. Si è visto peraltro che questi fenomeni investono l'intero Paese e non sono concentrati solo nel Sud, dove peraltro (non si può mettere la testa sotto la sabbia) il problema è aggravato dall'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche e - senza essere ipocriti - nella vita politica.

dopo Quatar, Botswana, Oman, Macau, Bhutan, Lituania, Namibia, Samoa, Cuba, a pari merito con l'Arabia Saudita. Noi siamo l'Italia! Nel 2009 - secondo il procuratore generale della Corte dei conti - è emerso un deciso aumento delle denunce per fatti di corruzione e concussione accertati, con un incremento fortissimo rispetto al 2008. Il numero delle denunce per fatti di corruzione e concussione accertati è fortemente aumentato rispetto all'anno precedente. Questa patologia chiama in causa la fragilità della società civile prima ancora che l'efficacia di controlli e sanzioni. Proprio per questo, tutti i contributi che vengono dalla società sono importanti e vanno valorizzati. il documento dei vescovi italiani su Chiesa e Mezzogiorno del febbraio scorso. I vescovi riconoscono che «tanti sembrano cedere alla tentazione di non parlare più del problema o di limitarsi a parlarne come di un male antico e invincibile»; invece vi è carenza di senso civico, una politica non credibile e quindi, sul piano socio-culturale, vi sono delle falle rilevantissime. Questa incultura evidente favorisce in alcune aree del Paese la criminalità organizzata e rischia di dettare i tempi e i ritmi della politica e dell'economia. Per mettersi a posto con la coscienza (vedo che il Governo è molto impegnato ad ascoltarci e comunque si è espresso in senso contrario), si afferma che la corruzione è un fenomeno fisiologico, radicalmente ineliminabile. Purtroppo però, quando la fisiologia diviene patologia, la Corte dei conti parla di una tassa occulta di 60 miliardi di euro l'anno: faremmo tutte le riforme economiche, verremmo incontro alle famiglie italiane e risolveremmo i problemi dell'occupazione! D'altronde, tra le principali ragioni che scoraggiano gli investimenti stranieri nel nostro Paese vi è proprio il livello di corruzione dilagante

Anche Confindustria ha ribadito che il ritorno alla legalità è l'unico modo per avere un'economia che continui a crescere; quindi, invitiamo Confindustria ad estendere il codice etico che ha applicato nelle Regioni meridionali a tutto il resto del Paese. motivo il Governo non è credibile? Il Governo in tema corruttivo non è credibile perché vi sono Ministri che sono indagati per corruzione. Voglio ricordare a tutti la corruzione in atti giudiziari che ha visto coinvolto direttamente o indirettamente il Presidente del Consiglio dei ministri. Ricordo il caso Previti, ricordo il caso Mills. Coinvolgiamo tutte le opposizioni e, vivaddio, se c'è qualche lezione su cui riflettere la si prenda anche dalle opposizioni. A noi non interessa un Paese ai minimi termini, non interessa un Paese che scenda sempre più nella scala dei diritti. D'altra parte, mi sembra veramente buffo parlare di leggi

che il Paese si liberi da un modo devastante di amministrare la cosa pubblica, in cui spesso la burocrazia è

lo hanno in particolare richiamato nel 2003. Sono stati fatti passi avanti, ma sicuramente non definitivi e risolutivi, ed anche il disegno di legge di cui si parla in questi giorni - e anche in queste mozioni, come quella da noi presentata - fatto dal Governo all'inizio di marzo è un ulteriore punto importante di discussione e risoluzione di questi problemi, che devono vedere chiaramente un lavoro *in* *progress* con continuità e determinazione.

una serie di misure per la trasparenza degli appalti pubblici, un complesso di interventi di riforma del controllo degli enti locali e l'inasprimento delle pene per i reati di corruzione, oltre ad alcune disposizioni riguardanti l'incandidabilità delle persone ai pubblici esercizi. La proposta di istituire un Piano nazionale anticorruzione e un Osservatorio sulla corruzione presso il Dipartimento della funzione pubblica corrisponde alla necessità di ricostituire organi e procedure della politica anticorruzione, colmando una carenza fermamente denunciata dal Rapporto ispettivo sul nostro Paese elaborato nell'autunno del 2009 dal Gruppo di Stati europei contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa.

Con questo disegno di legge, che prevede anche la soppressione del preesistente commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione,

siamo perfettamente d'accordo debba avvenire in maniera *bypartisan* - di quella che dovrebbe essere una seria politica contro la corruzione. mi basti ricordare la roboante dichiarazione nel gennaio del 2008

ha enfatizzato questo accordo come garanzia di sicurezza e trasparenza, al fine anche di impedire questa corruzione nelle pubbliche amministrazioni, specialmente in quella zona.

tutte le misure sulla trasparenza e l'attività amministrativa, sulle quali siamo assolutamente tutti concordi e sulle quali dobbiamo impegnarci per far sì che siano princìpi sempre più applicati e non rimangano soltanto norme su carta scritta. modo sono importanti le previsioni sui contratti pubblici, sulle quali ovviamente la trasparenza deve essere un principio sempre più applicato in maniera reale e non solo formale.

che potrebbe essere trasformata da sanzione accessoria a pena principale; l'introduzione di meccanismi premiali che incentivino la rottura del sodalizio tra corrotto e corruttore; la protezione dei dipendenti pubblici onesti che hanno il coraggio di denunciare i fatti corruttivi

ci siamo meravigliati che su alcune questioni non abbiamo avuto la possibilità di avviare un confronto, anche se il rappresentante del Ministero

sull'estensione del regime della confisca ai proventi accertati della corruzione e sull'annullamento dei benefici di legge nei reati di tipo economico e contro la pubblica amministrazione, non si riesca a trovare con la stessa maggioranza una convergenza. È difficile

nuova finestra"). Sono presenti in tribuna gli studenti del Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Trento, ai quali rivolgiamo il nostro saluto e l'augurio per le loro attività di studio. Signor Presidente, perché il dibattito parlamentare in cui siamo impegnati non venga immediatamente archiviato al momento stesso della sua conclusione e non lasci quindi il tempo che trova, è necessario che esso rappresenti il primo atto di una ripresa del dibattito pubblico sul fenomeno della corruzione, al fine di individuare le caratteristiche e la natura del fenomeno stesso e, soprattutto, di predisporre concrete, realistiche e immediate misure di contrasto. Si è preferito in questi mesi confinare il problema all'ambito giudiziario o genericamente pontificare contro la ricorrente e permanente corruzione della politica o peggio, come ha fatto il Governo, annunciare roboanti provvedimenti ai quali non si fa seguire nemmeno la presentazione delle proposte al Parlamento. È passato un mese da quel 1° marzo in cui il Consiglio dei ministri ha licenziato una semplice copertina, e delle due l'una, sottosegretario Alberti o quella era una pura operazione mediatica oppure le divisioni all'interno della maggioranza sono incomponibili su un tema così delicato come quello della corruzione. Tanto più sono roboanti e generici gli annunci, tanto meglio si prestano a sollevare polveroni che servono solo a coprire il mantenimento dello *status quo*. Il campo va sgomberato da due pregiudizi. In primo luogo, che si sia in presenza ancora oggi di una normale e fisiologica quantità di corruzione che caratterizza i sistemi politici e istituzionali dei Paesi più avanzati. In quest'ottica, secondo tale criterio, l'Italia sarebbe assolutamente in linea con gli altri Paesi e la corruzione non rappresenterebbe altro che un elemento di lubrificazione del rapporto tra affari e pubblica amministrazione, una componente che, se mantenuta in un ambito fisiologico, può addirittura rappresentare, secondo una teoria che ebbe un certo seguito qualche decennio fa, uno stimolo positivo alla crescita economica. Per i sostenitori di questa tesi non ci sarebbe, insomma, nessuna anomalia italiana in questa materia. Analogamente credo vada abbattuto un altro pregiudizio: non è sufficiente oggi proporre un parallelo con la stagione di Tangentopoli e di Mani Pulite, quasi che fossimo in presenza del riemergere dello stesso fiume carsico. Bisogna piuttosto impegnarsi nel comprendere le caratteristiche nuove del fenomeno corruttivo, leggerne le matrici e i percorsi e individuare un'adeguata strategia di contrasto. la corruzione in Italia ha assunto caratteri strutturali, di larga pervasività e diffusione che non determinano soltanto una gravissima decadenza dell'etica pubblica, ma anche una pesante ipoteca sul tasso di sviluppo dell'economia e sulla sua complessiva capacità di competizione, un tema di fronte al quale l'insieme delle classi dirigenti, non solo quelle politiche, dovrebbe pienamente misurarsi. Infatti, dopo la stagione di Mani Pulite e del crollo della prima Repubblica, la corruzione è entrata in una sorta di confortevole cono d'ombra cui non solo non ha conosciuto alcuna attenuazione, ma anzi ha potuto cambiare il suo modo d'essere per estendere i suoi tentacoli. Dalla fine degli anni Novanta all'inizio degli anni 2000 il fenomeno corruttivo si rifonda su basi nuove e approfitta largamente di alcuni provvedimenti legislativi: la depenalizzazione del falso in bilancio, le procedure di assegnazione delle opere nella gestione delle cosiddette emergenze, le varie edizioni dello scudo fiscale. Trasparenza e tracciabilità, infatti, sono gli antidoti fondamentali, i prerequisiti per ogni azione vera, concreta, di contrasto alla corruzione. In questo modo la corruzione ridefinisce le sue forme organizzative, i suoi sistemi di stabile comunanza, come qualcuno li ha definiti, la sua fitta ragnatela di conflitti di interesse, un nuovo rapporto insomma tra affari, pubblica amministrazione e mondo delle istituzioni. Insisto un momento sul falso in bilancio, quasi come elemento simbolico, perché ritengo che quello sia stato uno strappo storico profondo, un abbassamento drammatico dell'etica degli affari - non soltanto dell'etica pubblica un incentivo insomma all'economia cattiva contro quella buona. La procedibilità a querela di parte - vale a dire dei creditori e degli azionisti cioè il sostanziale affossamento - detto in termini più concreti - del principio che ci sia un interesse pubblico, generale al buon funzionamento delle imprese e dei mercati, promuove anche una selezione avversa nel mondo delle professioni interne ed esterne all'impresa. Il fenomeno, insomma, non riguarda - come ieri è stato detto da qualcuno - solo le istituzioni e la pubblica amministrazione, nei termini di comportamenti scorretti, di malversazione e di illiceità. Lo hanno dimostrato ieri in maniera magistrale Gerardo D'Ambrosio e Silvia Della Monica. Se fosse così, il fenomeno sarebbe addirittura - diciamolo in questo Bisogna leggere invece del fenomeno corruttivo le sue interrelazioni e i suoi sistemi di comunanza, le intelaiature di potere e di scambio di favori e di denaro, le forme di protezione del mercato che vengono costruite e garantite. Non sono più i partiti, il sistema partitocratico - come fu appunto negli anni Ottanta fino all'esito di Tangentopoli - a tenere in mano le briglie e ad assegnare i ruoli, in un contesto fortemente centralizzato e controllato. Sono singoli imprenditori o gruppi di imprenditori, filiere di corruzione che, attraverso un'azione penetrante di condizionamento e di vero e proprio orientamento delle scelte pubbliche, si appropriano delle risorse e ne distribuiscono anche illecitamente i vantaggi. il pendolo si sposta decisamente in direzione del privato e della sua capacità di conformare ai suoi interessi i comportamenti dei decisori nella pubblica amministrazione. Più evidente appare oggi il nesso il nesso tra tasso di corruzione e capacità di crescita dell'economia di un Paese. Tanto è forte la pervasività del fenomeno, tanto minore è la capacità e l'attitudine allo sviluppo. In una economia globalizzata, i Paesi in cui la corruzione è estesa tendono ad esportare corruzione e a richiamare e ad importare capitali grigi e di dubbia provenienza. È il tono complessivo, etico e competitivo, di un sistema Paese che si indebolisce quando la qualità della normativa economica si fa lasca, permissiva, implicitamente collusiva tanto più oggi, quando il mondo avanzato punta ad una nuova regolamentazione di qualità e ad una forte iniezione di etica negli affari e nell'economia. E a livello interno - nel caso italiano - oltre ad una caduta della capacità competitiva, assistiamo anche ad una grave distorsione della concorrenza, perché ad ogni imprenditore amico degli amici che sa dispensare denaro, favori o massaggi di varia natura ne corrispondono 10, 100, 1.000 che non sono amici degli amici e che stanno tutto il giorno a sudare e a faticare in azienda, ma che non fanno parte di quei sistemi di stabile comunanza a cui prima facevo riferimento. La risposta, allora, deve essere, per noi del Partito Democratico, a questa altezza dei problemi. Nell'ordine del giorno che abbiamo sottoscritto con l'UDC, SVP, Io Sud e Autonomie viene individuata con puntigliosità una serie molto dettagliata di misure e provvedimenti efficaci, operando in una combinazione virtuosa tra adeguamento al vincolo esterno e iniziativa interna. Per vincolo esterno si intende il recepimento integrale della normativa comunitaria nei diversi ambiti riguardanti la pubblica amministrazione, l'affidamento delle opere e la fornitura di beni e servizi: in generale, il rapporto tra pubblica amministrazione e soggetti economici. Per vincolo esterno si intende ovviamente anche la ratifica e l'esecuzione delle Convenzioni internazionali sulla corruzione.

Certo, collega Benedetti Valentini, esiste un problema di clima generale e si avverte la necessità di uno scatto dello spirito pubblico, ma c'è bisogno anche di un vincolo di coerenza tra il dire e il fare: altrimenti è pura demagogia. interventi mirati, incisivi, emblematici anche sul terreno della provvista, come si usa dire. I fondi neri, la modica quantità per le false fatturazioni, il falso in bilancio, lo scudo fiscale: non è attraverso questi provvedimenti

sia le procedure (anche amministrative) e le responsabilità amministrative che il versante degli strumenti specifici, penali e procedurali, di lotta alla corruzione. C'è bisogno, quindi, signor Presidente, di una grande continuità dell'azione riformatrice e di una seria azione di verifica sull'efficacia delle misure che si adottano. Altro che annunci mediatici. Un impegno di grande lena che noi dall'opposizione intendiamo sviluppare pienamente.

*(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, è vero: probabilmente in quest'Aula è stata persa un'ottima occasione per un dialogo ma non c'è dubbio che, se questa occasione è stata perduta, ciò non è imputabile in alcun modo alla maggioranza, né tanto meno al Governo. Potremmo limitarci a dire, onorevoli colleghi, che non sono le mozioni lo strumento attraverso il quale, in modo puntiglioso e apparentemente dettagliato, si affrontano costruttivamente tematiche così delicate, a fronte soprattutto del fatto che tutti in Aula abbiamo la piena consapevolezza che è in corso di definitiva gestazione un articolato e complesso provvedimento governativo proprio sul tema specifico. Quindi, a maggior ragione, buon senso e, se vogliamo, ragioni di economia dal punto di vista dell'utilizzazione delle nostre risorse lavorative avrebbero dovuto indurre a finalizzare le mozioni ai portati di principio, sui quali ritengo tutti necessariamente si debba essere d'accordo. Invece, abbiamo dovuto prendere atto che tutte le mozioni presentate dall'opposizione - che, sì, per carità, come regolarmente avviene in situazioni di questo tipo, possono presentare anche un singolo punto astrattamente condivisibile si sono tradotte in una indiscriminata critica a tutta l'azione svolta dal Governo e dalla maggioranza in tema di giustizia e di contrasto alla criminalità e all'illegalità in tutte le sue forme, sia per ciò che è stato fatto sia per ciò che ci si accinge a fare. Onorevoli colleghi, le mozioni non possono essere prese per la parte che conviene e scartate per quella che non conviene nel momento stesso in cui ci si confronta. Dobbiamo valutare le mozioni nel loro complesso, nella loro portata, ma soprattutto nel filo conduttore che le anima, nello spirito che, in qualche modo, ne ha motivato la predisposizione e i contenuti, e nelle loro finalità. Allora, non v'è dubbio che in nessuna delle mozioni presentate dall'opposizione questa volontà costruttiva di dialogo emerge. Emerge, piuttosto, una critica indiscriminata e manichea a tutta l'azione che il Governo e la maggioranza hanno condotto e stanno conducendo. Azione che, una volta per tutte, cari colleghi, dovrete ammettere ha determinato nella lotta alla criminalità organizzata risultati mai visti nella storia di questo Paese. L'altro aspetto che credo parimenti non possa che indurre il Governo e la maggioranza ad assumere la posizione che hanno

che quanto oggi stiamo trattando non è certamente frutto di un'evoluzione genetica che improvvisamente, negli ultimi due anni, ha contraddistinto questo Paese: è un fenomeno che affonda le proprie radici lontano; un fenomeno che, se oggi ha le dimensioni che ha, sicuramente travolge e involge responsabilità che non sono soltanto di chi oggi ha la guida del Paese, che anzi risultati rilevanti, in un aspetto che non è trascurabile nella lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione - quello legato alla lotta alla criminalità organizzata - ha già significativamente dato. L'altro aspetto, che forse è quello più importante per il ruolo al quale assolviamo, è che la vostra continua a rimanere una visione assolutamente pessimistica e colpevolista della società; una visione che è inaccettabile, nel momento stesso in cui noi non dobbiamo dimenticare che il bene supremo che dobbiamo garantire è la libertà. E questo messaggio, per l'ennesima volta, i cittadini ve l'hanno dato, ma in quella sorta di deriva giustizialista, di furore manicheo-giacobino che continua a contraddistinguervi e a non farvi capire che di *maîtres à penser* gli italiani non ne vogliono sapere, voi riuscite a non capire che quello che il Governo e la maggioranza hanno già fatto in materia di giustizia i cittadini italiani lo approvano, lo hanno approvato e continueranno ad approvarlo. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Non è inasprendo inutilmente sanzioni e controlli che si combattono fenomeni come la criminalità organizzata e come la corruzione nella pubblica amministrazione: semmai, con un percorso etico, valoriale, completamente diverso, perché un inasprimento indiscriminato di misure inutilmente invasive è stato già bocciato ripetutamente dai cittadini italiani quando hanno espresso il loro consenso o il loro dissenso rispetto all'azione di governo. Ed allora, Ed allora, era questo lo spirito con il quale ci dovevamo confrontare: non cercare di tornare nuovamente su argomenti che, soprattutto in tema di giustizia, hanno già avuto la loro ampia trattazione, né tornare ancora a reinserire critiche che sapete perfettamente non essere fondate. Sono queste le ragioni per cui ritengo si sia perduta oggi una grande occasione di dialogo su un tema che non può che vederci tutti uniti,

Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

venisse accolta dal Governo. È una scelta politica, però significa, Presidente, alla fine, trasformare questa discussione nel seguito degli annunci dati in campagna elettorale dal Presidente del Consiglio

oltre a quella già dichiarata di votare distintamente sui documenti presentati, è di enucleare dal documento a mia prima firma, sottoscritto da diversi colleghi, due punti specifici.

chiedono di estendere ai proventi accertati della corruzione - inclusa quella politico-amministrativa - il regime della confisca

inviti rivolti al Governo al fine di focalizzare due aspetti estremamente pragmatici che il Governo dovrebbe impegnarsi ad inserire con proprie proposte nel corpo legislativo del nostro Paese.

sono contraria ad una votazione per parti separate. Stiamo infatti trattando una materia assai complessa e molti degli argomenti sviluppati nelle mozioni sono già stati da noi trattati con leggi recenti; altri, come la riforma più complessa del codice di procedura penale, sono oggetto di dibattito parlamentare e, quindi, di un confronto che si sta svolgendo svolgendo in Commissione giustizia.

Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni. Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento sarà posto ai voti l'ordine del giorno G1, anch'esso per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Colleghi, per favore, due non fanno uno e tre non fanno due. è veramente umiliante per la Presidenza assistere a queste scene.

**Il Senato non approva.**

*(PdL)*. Signor Presidente, signori senatori, rappresentanti del Governo... Mi consenta un attimo di pausa, chi intende uscire lo faccia rapidamente. Consentiamo senza indugiare troppo al senatore Possa di illustrare la sua mozione. Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Presidente. La mozione che mi accingo ad illustrare - che ha come primo firmatario il presidente D'Alì, che interverrà fra un momento per alcune precisazioni - ha per oggetto la politica del nostro Governo sulla complessa questione del riscaldamento globale, e ne chiede un profondo riorientamento dopo il sostanziale fallimento della Conferenza COP tenutasi a Copenaghen lo scorso dicembre. Desidero sottolineare in premessa che condividiamo pienamente l'esigenza di una maggiore sostenibilità energetica della nostra società, nonché l'esigenza di tutela del clima, bene fondamentale dell'ambiente in cui viviamo. Tuttavia, la linea politica assunta in questi anni sul problema dei cambiamenti climatici dall'Unione europea ci pare molto criticabile su punti di grande importanza. La mozione ha come punto di partenza una valutazione nettamente negativa a riguardo delle analisi climatiche presentate in questi anni dall'IPCC, il noto organismo afferente all'ONU. Non convince affatto, per l'insufficiente fondamento scientifico, l'attribuzione fatta dall'IPCC, praticamente senza incertezze, all'anidride carbonica da combustione dei combustibili fossili della causa del riscaldamento dell'atmosfera, peraltro modesto, osservato negli ultimi due secoli. L'IPCC non tiene in debito conto che nella dinamica straordinariamente complessa del sistema atmosfera-oceani-terre emerse vari importanti processi sono a tutt'oggi poco conosciuti. Tra essi, ad esempio, i processi di formazione delle nuvole, le diverse azioni energetiche esercitate dai vari tipi di nuvole, i comportamenti fisici e chimici del vapore acqueo e dei gas serra nei diversi strati dell'atmosfera, gli effetti climatici dei vari tipi di aerosol che possono trovarsi nell'atmosfera. Ancora meno convincenti sono le previsioni dell'IPCC riguardanti l'evoluzione del clima terrestre nei prossimi decenni fino alla fine del secolo. Ciò sia per l'inadeguata conoscenza della base fisica del clima sopra sottolineata, sia per la grande complessità delle interazioni energetiche che hanno luogo alla superficie della Terra e per la conseguente estrema difficoltà della loro modellizzazione matematica. In particolare sono affette da errori difficili da valutare le previsioni degli aumenti di temperatura dell'atmosfera, delle variazioni di piovosità e dell'aumento del livello degli oceani, anche se effettuate mediante i modelli matematici estremamente sofisticati ultimamente sviluppati. Su queste serie incertezze previsionali purtroppo l'IPCC sorvola. Assolutamente non condivisibili sono infine le drammatiche previsioni fatte dall'IPCC a riguardo delle conseguenze economiche e sociali dei cambiamenti climatici previsti. L'IPCC sottostima gravemente le formidabili capacità di adattamento dell'uomo alle più diverse condizioni ambientali. In particolare non condivisibili sono le stime dei futuri danni dovuti all'assenza di un'immediata drastica riduzione dell'immissione di anidride carbonica nell'atmosfera e le stime dei costi (attuali) di tale riduzione. II *modus operandi* dell'IPCC sta ora sollevando anche varie altre pesanti critiche, come evidenzia bene il recentissimo libro «*L'imposture climatique*», di Claude Allègre, ex ministro del Governo Jospin. In sostanza l'IPCC risulta completamente controllato da un ristretto gruppo di alcune decine di scienziati e funzionari ispirati da ideologie verdi radicali, che agisce con modalità totalitarie, eliminando ogni voce non allineata (interna ed esterna). Inoltre, ultimamente due scandali hanno gettato una luce negativa sull'IPCC. Alcuni *hacker* hanno scoperto che Phil Jones, personaggio importante dell'IPCC, direttore dello Hadley Center dell'università inglese East Anglia, su cui l'IPCC si basa per il delicato calcolo della temperatura media mondiale annuale dell'atmosfera al suolo, ha inviato a più riprese ai corrispondenti che gli forniscono i dati per tale calcolo *e-mail* richiedenti l'eliminazione delle misure di temperatura non congruenti con la teoria del riscaldamento globale. Lo scandalo ha costretto Jones alle dimissioni. Un altro scandalo ha riguardato il direttore dell'IPCC Pachauri, che un'inchiesta giornalistica ha rivelato essere un affarista impegnato nel *business* delle energie rinnovabili, *business* d'altra parte fortemente promosso dall'IPCC. Il poco tempo a disposizione consente solo una succinta critica della discutibilissima politica dell'Unione europea riguardante la questione del riscaldamento globale, una politica radicale, costosa, perseguita con velleità di primazia mondiale, dogmaticamente allineata senza incertezze alle indicazioni dell'IPCC, spesso ancora più catastrofista di tali indicazioni (come mostra il frequente riferimento al rapporto Stern), con limitatissimi effetti sul clima. Il primo importante atto di tale politica è stata la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto con l'impegno ad una riduzione dell'8 per cento (rispetto al 1990) delle emissioni di gas serra antropogenici da conseguire negli anni 2008-2012. Nessun altro Paese firmatario del Protocollo ha sottoscritto un impegno così gravoso. L'Italia, con il ministro verde Edo Ronchi, ha convenuto una riduzione del 6,5 per cento, che penalizza ingiustamente il nostro Paese. I risultati del Protocollo di Kyoto sono ormai evidenti. A fronte di una modestissima riduzione dell'emissione di anidride carbonica da combustione, praticamente senza effetto sul clima, si riscontrano: sviluppo di pesanti burocrazie europee e nazionali per controllare le emissioni degli impianti, distorsioni della concorrenza nel mercato europeo dell'energia causate dagli aiuti di Stato consentiti per le fonti rinnovabili, blocco dell'incremento dell'utilizzazione del carbone, aumento del costo dell'energia elettrica, sviluppo dell'industria assistita delle fonti rinnovabili, delocalizzazione di impianti energivori, perdita di competitività. Per inciso, il conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 6,5 per cento appena ricordato è stato possibile nel nostro Paese negli anni 2008 e 2009 solo per effetto della grave crisi finanziaria ed economica mondiale in via di superamento. La seconda e ben più radicale decisione dell'Unione europea è stata l'Accordo 20-20-20 sottoscritto dai ventisette Paesi dell'Unione nel marzo del 2007. Gli obiettivi "vincolanti" da raggiungere entro il 2020 per via di tale accordo sono molto gravosi. Tale unilaterale assunzione di pesanti impegni da parte dell'Unione europea è frutto dell'ambizione a svolgere un ruolo di primattore sulla scena mondiale, ambizione che le vicende del COP 15 hanno dimostrato priva di realismo. Lo sforzo per il conseguimento di questi obiettivi determinerà un pesante aggravamento delle conseguenze negative sopra elencate prodotte dal Protocollo di Kyoto. I benefici ambientali saranno molto modesti, data la limitatezza della quota di anidride carbonica emessa dall'Unione europea rispetto al totale mondiale. Ma questa radicale politica dell'Unione europea a riguardo del riscaldamento globale sta determinando un effetto ben più grave, cari colleghi. Il totale dogmatico appiattimento sulle tesi catastrofiste dell'IPCC, senza lasciar spazio ad alcuna critica, il rilevante appesantimento burocratico indispensabile per la verifica del conseguimento degli obiettivi vincolanti e la volontà di controllare dirigisticamente e tecnocraticamente tutte le produzioni, onde promuoverne l'ecocompatibilità, tendono ormai a connotare l'intera azione dell'Unione in termini *post* democratici. È anche importante sottolineare che sussiste un'obiettiva grande difficoltà a realizzare urgentemente in tutti i Paesi una qualche forma di limitazione della combustione dei combustibili fossili (come sarebbe indispensabile se fosse vera l'ipotesi che l'aumento della temperatura dell'atmosfera sia dovuto all'aumento della concentrazione di anidride carbonica). Non si vede perché i grandi Paesi emergenti come Cina, India e Brasile, che hanno ancora emissioni *pro capite* molto inferiori a quelle dei Paesi sviluppati, debbano penalizzare il loro sviluppo limitando l'uso del carbone. Questi Paesi non sottoscriveranno mai impegni a limitazioni delle loro emissioni tipo «*cap and trade».* (molto onerosi) ai Paesi in via di sviluppo che si stanno prospettando nei Paesi sviluppati a titolo di assistenza nella lotta ai cambiamenti climatici non potranno mai raggiungere il livello di appetibilità richiesto. In base alle considerazioni critiche sommariamente riassunte, la mozione chiede al Governo di intervenire presso l'Unione europea per ottenere un profondo riesame della politica sul riscaldamento globale, avvalendosi in particolare della clausola di revisione dell'Accordo 20-20-20 ottenuta dal presidente Silvio Berlusconi nel Consiglio europeo del dicembre 2008 al momento della firma del *Burden Sharing Agreement* per tale Accordo. In particolare la mozione chiede al Governo di adoperarsi presso l'Unione europea per la revisione della *governance* degli organi preposti in sede ONU alla determinazione delle strategie ambientali, con l'avvicendamento del dottor Pachauri e del commissario De Boer; una profonda riorganizzazione dell'IPCC per riportare alla massima priorità

sulla scienza e non sulle diagnosi e previsioni altamente ideologizzate dell'IPCC e in modo da orientarla verso accordi internazionali di contenimento dei consumi energetici che siano rispettosi delle esigenze di sviluppo dei Paesi emergenti; l'ulteriore promozione in sede internazionale di attività di ricerca sul tema dei cambiamenti climatici, anche con esplicito riferimento all'area euromediterranea.

onorevoli senatori, noto che il Governo è assente. La mozione n. 260, presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori, impegna il Governo, che non vedo, a dare piena attuazione agli impegni assunti nel dicembre 2009 sulle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, muovendosi coerentemente con quanto è stato deciso in sede di Unione europea. Riteniamo infatti, alla vigilia degli incontri internazionali di Bonn, che sia importante per l'Italia mantenere un efficace coordinamento ed una positiva interazione con i *partner* comunitari nello sviluppo di iniziative. indipendentemente da quanto ciascun Paese può fare da solo ed in via autonoma, ed è certamente molto, queste iniziative hanno più successo ed efficacia se sono inquadrate in un contesto continentale organizzato. L'impegno che chiediamo al Governo di assumere, consistente nel mantenere ed onorare gli impegni già sottoscritti dall'Italia in tutte le sedi internazionali e comunitarie riguardanti i cambiamenti climatici e la protezione dell'ambiente, si inquadra perfettamente in una linea che, indipendentemente dal colore dei Governi e delle coalizioni (coalizioni e Governi che si sono succeduti nel tempo), accomuna tutte le parti nella volontà di promuovere l'implementazione e, ove necessario, il miglioramento degli accordi di Copenaghen, con particolare riferimento ad alcune lacune che si sono evidenziate nei meccanismi negoziali del *Summit* del COP 15 ed ai passi ancora da compiere per la definizione e la verifica di obiettivi ulteriori. È questa la linea seguita fin qui da tutti i Governi italiani, dai Governi europei in generale e dalla maggioranza dei Paesi che nel tempo, nelle diverse sedi negoziali internazionali, da molti anni riconoscono l'importanza della questione climatica e delle sue implicazioni socio-economiche, oltre che strettamente ambientali. Affrontare la sfida piuttosto che attardarsi a negarla è un'occasione importante per l'economia italiana e per il nostro sistema produttivo; un'occasione di crescita e innovazione per la quale chiediamo al Governo di valorizzare le eccellenze dell'industria e della ricerca nazionale nell'innovazione ambientale, anche definendo agevolazioni stabili per impianti che producono o che utilizzano fonti rinnovabili pulite, in modo da superare le ricorrenti incertezze e l'alternare degli incentivi di volta in volta promessi. Il risparmio e l'efficienza energetici, compresa l'efficienza delle reti, sono i punti essenziali, insieme alla promozione delle fonti rinnovabili, per una politica di impegni che vede l'Italia muoversi insieme agli altri grandi Paesi industrializzati e all'Unione europea. Sono questi gli impegni della nostra mozione. Sono questi gli impegni in vista dei passi ulteriori che il negoziato sul clima deve compiere nel 2010 e nel 2011. Se l'Accordo di Copenaghen è stato per certi versi deludente, esso ha tuttavia coinvolto per la prima volta Stati Uniti, Giappone, Brasile, Sudafrica, India e Cina, Paesi che rendono conto quasi dei quattro quinti delle emissioni mondiali derivanti dall'utilizzo di energia. L'Unione europea, e l'Italia in essa, ha presentato formale adesione all'accordo il 28 gennaio 2010, indicando obiettivi di riduzione non inferiore al 20 per cento, che la mozione di maggioranza finge di non ricordare. Con riferimento alla stesura di trattati legalmente vincolanti con meccanismi di verifica e sanzioni la trattativa su tempi e scadenze non è comunque chiusa ed è anzi dato per scontato che, al più tardi nel 2011, questo obiettivo sarà raggiunto. Da ultimo, il Consiglio europeo del 16 marzo ha preso impegni chiari sulla tutela dell'agricoltura e delle biodiversità rispetto alle conseguenze dei cambiamenti climatici. In quella, come in tutte le altri sedi negoziali, l'Italia era comunque presente ed il Governo italiano - e stiamo parlando di quello attuale - ha preso impegni chiari. Per questo sorprende sinceramente leggere ancora una volta una mozione di alcuni esponenti della maggioranza che nega il problema e mette in dubbio la credibilità di chi ha sottoscritto gli accordi e gli impegni, gettando nell'imbarazzo quello stesso Governo che dice di sostenere. Ricordiamo che, esattamente un anno fa, nel corso di un'imbarazzante seduta del Senato, il Governo ha dovuto chiedere alla sua maggioranza di riscrivere per ben tre volte la mozione sul clima in vista del G8 e del COP 15 di Copenaghen. Per questo si resta stupefatti nel leggere un atto di impegno in cui si dice che «l'Italia ha assunto obbiettivi ed oneri estremamente penalizzanti» e che «l'Unione europea in materia ambientale ha adottato senza la minima incertezza le tesi catastrofiste basate sui contenuti dei rapporti ONU-IPCC e di alcuni studiosi inglesi alle quali gli altri Governi si sono acriticamente accodati». Si insultano così in un solo colpo l'Unione europea (di cui siamo parte), l'ONU (di cui siamo parte) e tutti i Governi; colpisce l'uso delle parole e la terminologia piuttosto leggera, se non sconveniente, che viene adoperata in questo testo. Si arriva ad impegnare il Governo italiano a fare qualcosa di assolutamente irrituale, vale a dire «promuovere in sede ONU la revisione degli assetti degli organi preposti alle determinazioni delle strategie ambientali» mediante una deliberazione del Senato italiano volta ad ottenere la rimozione del presidente dell'IPCC e del Commissario per il clima dell'ONU, dichiarando il primo «manifestamente (...) fazioso e inaffidabile» (così si legge nella mozione), mentre il secondo sarebbe poco capace perché non segue la scala di priorità indicata dai firmatari della mozione. il commissario De Boer ha riconosciuto di non aver saputo o potuto raggiungere un accordo migliore di quello di Copenaghen e per questo, dal 1° luglio, lascerà il suo incarico, dal quale non va pertanto dimissionato dal nessun Governo, tantomeno dal Senato italiano. Le stesse critiche, opinabili ma legittime, si sarebbero potute esprimere in un linguaggio più corretto e adeguato ai rapporti internazionali. Non si comprende peraltro come il Parlamento italiano possa dichiarare decaduto il cosiddetto Accordo 20-20-20 raggiunto in sede europea. Un conto è avvalersi di una clausola, ben altra cosa è la denuncia unilaterale di un accordo tra più parti. Sappiamo che il Governo è scettico sull'obiettivo del 30 per cento di riduzione, ma rinunciare anche a quello del 20 per cento significa porsi fuori dai negoziati. La mozione di maggioranza addirittura dichiara «gravosissimi» gli impegni connessi con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e, subito dopo, riprendendo un linguaggio assolutamente inaccettabile, chiede al Governo italiano di «adoperarsi affinché la politica ambientale dell'Unione europea abbandoni la linea sinora imposta» dagli inglesi e dai tedeschi. Per quanto approssimativa possa essere la conoscenza dell'italiano, il modo di esprimersi non è mai casuale. Quando si chiede di abbandonare inglesi e tedeschi ci si riferisce ai popoli interi oppure ai soli Governi che il Governo italiano ritiene invece *partner* affidabili e stretti alleati? A quali posizioni ci si riferisce? La politica estera italiana negli ultimi tempi è piuttosto singolare, ma, addirittura, nella mozione si chiede di sconfessare tutti i Commissari europei all'ambiente succedutisi nel tempo; tutti quanti, dal primo a quello in carica, il quale dovrebbe evidentemente fare le valigie. La mozione n. 248 rileva infine che la linea dettata dal Senato in sede di esame di specifiche mozioni sul clima non risulta essere stata adeguatamente seguita in occasione di molti incontri internazionali;

Del tutto illogico, e probabilmente contrario ad ogni *standard* tecnico di redazione di atti d'indirizzo di politica internazionale, è l'impegno che il Governo dovrebbe assumere per sospendere non meglio precisati progetti internazionali, con ciò minando definitivamente l'affidabilità e la credibilità del nostro Governo. Dal 2005 in Italia si sono intensificate le misure che puntano ad una riduzione delle emissioni, come per esempio l'incentivazione alle fonti rinnovabili e gli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi, che danno benefici anche per la competitività dell'industria nazionale. Questi sono gli obiettivi europei che noi dell'Italia dei Valori chiediamo al Governo di confermare e fare propri. Sono presenti in tribuna gli studenti del liceo classico «XXV Aprile» di Portogruaro, in provincia di Venezia. Rivolgiamo loro il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio.

la mozione n. 262 è un tentativo per evitare al nostro Paese e a questo Senato di fare un'ennesima figuraccia a livello internazionale. perché oggi la maggioranza propone una mozione che cercherò di spiegare essere inapplicabile da qualsiasi Governo, ed è quella stessa maggioranza che pochi mesi fa ci ha fatto votare una mozione che - ahimè - ha reso ridicolo il Paese, ed anche questa autorevole istituzione, agli occhi del mondo. Era infatti l'unica mozione, a mia conoscenza, in cui un Parlamento a livello mondiale

evitare questa abitudine di votare mozioni che poi lasciano il tempo che trovano e cercare invece, ove possibile, di approvare mozioni che abbiano un senso, che scientificamente abbiano

chiedono al Governo di non tener conto (ed anzi, di impugnarlo con una certa fantomatica clausola Berlusconi, che non esiste) dell'impegno che lo stesso nostro Governo ha preso a livello europeo di onorare quello che passa sotto il nome di Accordo 20-20-20,

non solo è pronta a conseguire quegli obiettivi che in base all'Accordo 20-20-20 sono per essa anche più stringenti di quelli che dovremmo raggiungere in Italia, ma ha già dichiarato che andrà oltre quegli stessi obiettivi,

a chi propone gli impegni più stringenti di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, perché vogliono marciare il più rapidamente possibile - laburisti e conservatori - verso una società che impieghi meno fonti fossili possibili. Pertanto, siamo al paradosso per cui la maggioranza di centro-destra si conferma come l'unica forza politica - ahimè - a livello mondiale

a Copenaghen, luogo in cui non è stato raggiunto un accordo vincolante per tutti i Paesi per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, si sia però verificato un fatto straordinario,

seppur diversi e forse non adeguati alla sfida in atto, comunque tutti volti a ridurre le emissioni di anidride carbonica puntando sulle fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica e sulla riduzione del ricorso alle fonti fossili.

in Italia questa non è la migliore stagione politica dell'ambientalismo; d'altro canto, la funzione cui è ridotto il Ministero dell'ambiente è nota a tutti.

alle sue spalle: finalmente escono allo scoperto i negazionisti del centrodestra. Non siamo di fronte ai cosiddetti climascettici, né

a spiegare che in fondo i Paesi che hanno o avranno in prospettiva maggiori emissioni sono in fondo i nostri competitori extraeuropei (gli statunitensi, i cinesi, gli indiani, i messicani, i brasiliani, i sudafricani),

l'Europa a quel tempo scenderà al 30 per cento, mentre i Paesi asiatici ci supereranno. Tra un po', del resto, la Cina supererà gli Stati Uniti tra i Paesi energivori e anche emettitori.

Di fatto, l'emissione di anidride carbonica dovuta a questo aumento di energia sarà superiore al 57 per cento. L'impatto di questo aumento sul riscaldamento globale sarà drammatico da sé, anche se fosse una causa aggiuntiva, in particolare nelle aree aride e semiaride del pianeta. D'altro canto su siccità,

L'aumento medio della temperatura - altro che 2 gradi centigradi, come citiamo nella nostra mozione - entro la fine del secolo sarà di almeno 4 gradi centigradi, con un innalzamento degli oceani di 60 centimetri con conseguenze devastanti sugli ecosistemi, sulle scorte di acqua e sugli insediamenti umani. Questo è sinteticamente il quadro condiviso da tutta la comunità scientifica e politica.

È evidente che questa è esattamente la tesi dei "clima-scettici". In fondo questa è la tesi: l'emissione dell'anidride carbonica è solo una concausa dell'innalzamento del riscaldamento globale. Ma nella vostra mozione siamo in presenza di una aggravante in più. essa si nega l'evidenza e la conclusione sta tutta dentro una logica che pervade in qualche modo l'azione complessiva di questo Governo. Ogni Paese - questa è la logica - si arrangi da sé, così come ogni territorio del nostro Paese; ogni individuo si arrangi da sé senza regole, senza impegni, senza responsabilità né verso gli altri né verso il futuro. Il verbo di fondo che sta alla base del blocco sociale al quale vi riferite è sempre lo stesso, ed è facile: è quel consumare, consumare, consumare. consumare, consumare. Magari qualcuno di voi si atteggia, si attrezza e fa la critica al mercatismo. Ma anche questa nozione è declinata nella vostra mozione con gli occhiali del consumismo più sfrenato e senza remore di alcuna natura. Per questo motivo presentiamo una nostra mozione che segni la differenza. Rispetto ai temi che interrogano il futuro, non possiamo comportarci da irresponsabili, da attori mossi dal copione di un consumismo sfrenato. Sappiamo anche che non serviranno richiami etici e culturali legati alle tradizioni non solo culturali ma anche culturali ma anche politiche, all'ispirazione dei cattolici democratici, dei riformisti, degli ecologisti e neanche a quella dei liberali. Allora l'invito è di confrontarci facendo alcuni conti

Sappiamo dare risposte, tra l'altro, alle esigenze di nuova energia stabile e sicura, perché parliamo dei nuovi diritti applicati a quei Paesi che si sono aperti al mercato, che sono usciti da una economia chiusa. Tra questi, cito il diritto all'accesso all'energia. Insomma, esemplificando il contenuto della nostra mozione: vorremmo spingerci a parlare insieme di *green economy*, un grande piano mondiale di investimenti in energia pulita da estendere ai Paesi in via di sviluppo e che deve essere finanziato dai Paesi già sviluppati.

in questo modo si capisce qual è la discussione che si può sviluppare. In sostanza, nella nostra mozione si rileva efficienza energetica, un *mix* intelligente di fondi energetici, ricerca ed innovazione, diffusione delle tecnologie a livello globale, stimoli economici e fiscali, interventi sulle reti, sostegno al piano solare del Mediterraneo, difesa delle foreste, tutela della biodiversità e Questa è la nostra mozione. Per votarla, però, è necessario un pre-requisito: bisogna avere fiducia nel futuro e non avere - sempre e comunque - la necessità di solleticare le paure,

senatori, è ormai dimostrato il rapporto di causa-effetto tra l'operato dell'uomo e i cambiamenti climatici. Ricollegabili ad esso sono: l'aumento medio del livello del mare su scale globale, il ritiro dei ghiacciai, l'estremizzarsi delle precipitazioni in alcune aree, la desertificazione di altre aree del pianeta. Questo ultimo processo naturalmente interessa anche il territorio italiano. Considerando le innegabili conseguenze dei cambiamenti climatici, si sono intensificati negli ultimi anni i vertici mondiali sul clima: vertici nei quali viene richiesto ai Governi una presa di coscienza della gravità del problema e, soprattutto, un impegno concreto.

di piani attuativi per gli obiettivi preposti, come nel caso della Conferenza sul clima tenutasi a Copenaghen lo scorso dicembre: questo è un punto su cui mi soffermerò fra poco. Prima, però, credo sia doveroso sottolineare che, sia la Conferenza di Copenaghen, sia le conclusioni dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* - la cui essenza è rimasta la stessa da 20 anni a questa parte - hanno avuto il merito di confermare che le attività umane, immettendo sempre più gas a effetto serra nell'atmosfera, stanno davvero alterando il clima. È una considerazione tutt'altro che scontata, non soltanto perché è al centro di un concitato dibattito scientifico, ma anche perché è una questione che ancora oggi molti Governi tendono a minimizzare. Questi rapporti, inoltre, rivestono una grande importanza in quanto base delle risoluzioni dell'ONU, del G8 e dell'Unione europea in ordine alle politiche ambientali e in quanto sono, in particolare, alla base di accordi impegnativi.

dovuto procedere ad una revisione del cosiddetto Accordo del 20-20-20, a suo tempo stipulato solamente dagli Stati europei, come già avvenne per il Protocollo di Kyoto.

non crediamo sia giusto chiederne lo scioglimento e riteniamo, anzi, indispensabile prendere in considerazione ogni possibile rivisitazione, al fine di fare aderire all'accordo anche i Paesi maggiormente inquinanti

ad esplicitare la volontà di perseguire le politiche climatiche in modo autonomo e non vincolante in sede internazionale. Per coinvolgere quanti più Stati possibili, pensiamo si debba procedere

Invitiamo il Governo a non criticare in modo sterile il Protocollo di Kyoto e l'Accordo 20-20-20 anche perché in questo modo si espone solo l'Italia al rischio di apparire incapace di comprendere il problema ambientale nella sua complessità e gravità. Oggi, invece, siamo tutti consapevoli del fatto che l'inquinamento, come l'inflazione, è una tassa subdola che colpisce soprattutto la popolazione, anche se in modo indiretto; pertanto, non si può più rimandare. Sebbene il problema principale non sia certo quello dell'immagine del nostro Paese all'estero, non si può far a meno di pensare che di mezzo c'è anche la credibilità della politica italiana. Queste sono soltanto alcune delle ragioni per cui il Governo dovrebbe rivisitare gli impegni di riduzione delle emissioni di CO2 su livelli per l'Italia più equilibrati rispetto a quelli assunti dagli altri Stati membri aderenti. A nostro avviso, l'Italia potrebbe svolgere un ruolo da protagonista, impegnandosi in tutte le sedi diplomatiche ed istituzionali al fine di farsi promotore di una intesa che coinvolga i maggiori Paesi inquinanti, sostenendo anche una condivisione degli impegni connessi con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili mediante uno sviluppo dei mercati internazionali delle emissioni. Voglio concludere con una frase pronunciata dal responsabile dimissionario del segretariato ONU sul clima, Yvo de «La via per affrontare il cambiamento climatico è lunga e per raggiungere la perfezione ci vuole molta pratica». Chiaramente, queste parole sono soprattutto un invito; un invito che accogliamo mettendoci immediatamente al lavoro in questa direzione.

Signora Presidente, come ha preannunciato il presidente Possa, intervengo solamente per alcune precisazioni dovute al fatto che la nostra mozione è stata presentata il 25 febbraio 2010 nel frattempo, sono intervenuti alcuni fatti importanti che ne confermano in pieno i contenuti e le proposte. In particolare: l'ONU ha avviato un'indagine ispettiva sull'operato della IPCC; Yvo de Boer, commissario della Convenzione ONU per il cambiamento climatico, si è dimesso e non sarà più commissario dal 1° luglio di questo anno, così come chiedevamo nel nostro dispositivo; al vertice italo-francese il Presidente del Consiglio ha avviato l'interlocuzione, assieme al presidente Sarkozy, proprio sull'accordo del 20-20-20 e come prima mossa, ne ha escluso ogni possibile modifica a rialzo. In conseguenza di ciò, ho predisposto alcune varianti al testo della mozione, nella parte degli impegni, che mi permetto di trasmettere alla Presidenza perché ne possa dare conto al Governo ed ai colleghi.

sui rischi ed i pericoli cui è sottoposto il pianeta a causa del cosiddetto riscaldamento globale. Senz'altro alcuni fatti, come l'aumento della temperatura del Mar Mediterraneo dell'estate scorsa, il conseguente aumento delle precipitazioni nel nostro Paese questo inverno, che ha provocato frane e purtroppo vittime umane, lo scioglimento dei ghiacciai rappresentano dati inconfutabili che evidenziano un cambiamento climatico in atto che non bisogna assolutamente sottovalutare. Ma quanta influenza ha l'uomo su tale cambiamento climatico? Le più recenti valutazioni degli esperti sulla situazione mondiale del clima dimostrano che gli annunci catastrofici di qualche mese fa non sono confermati da dati scientifici. I rapporti dell'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) sul cosiddetto riscaldamento globale che in questi ultimi anni hanno prodotto le basi delle risoluzioni dell'ONU, del G8 e dell'Unione europea in tema di politiche ambientali si sono dimostrati inaffidabili. Eppure, sulla base di tali rapporti è stata fondata la stessa ossatura degli impegni straordinariamente pesanti presi dall'Unione europea. Mi riferisco soprattutto all'Accordo del 20-20-20. Nell'ambito di tali accordi l'Italia ha assunto obbiettivi ed oneri estremamente penalizzanti e, se le analisi effettuate fino ad oggi si rivelano errate, è evidente che occorre un cambiamento sostanziale della politica di intervento. In altre parole, occorre ripensare le strategie per la mitigazione del rischio. Fino ad oggi è prevalsa l'opinione comune generale che bisogna affrontare una serie di costi nel presente per evitare i rischi futuri, ma in questo modo ogni Stato e, all'interno di ciascuno Stato, ogni settore economico, cerca di pagare il meno possibile, cerca di sopportare il minor peso possibile dell'intervento complessivo, con la conseguenza che, purtroppo, tutto si blocca. Senz'altro questa concezione della strategia di intervento ha contribuito al fallimento del Vertice di Copenaghen. In tale sede, l'Italia ha affermato la necessità di assumere impegni in ordine alla riduzione delle emissioni che risultino vincolanti per tutti i Paesi e confrontabili tra di loro. In particolare, l'Italia ha chiesto, giustamente, che anche gli Stati Uniti riducano le emissioni con obiettivi paragonabili a quelli europei, dal momento che l'Europa si è autonomamente impegnata a ridurre le emissioni del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Ma se gli Stati Uniti e la Cina, che da soli producono la metà dei gas serra di tutto il pianeta, non hanno voluto assumere impegni per la riduzione del CO2 con caratteristiche vincolanti, come è possibile pensare di continuare da soli una battaglia che peraltro viene fondata su dati catastrofici che si rivelano addirittura errati? È chiaro che la posizione più equilibrata è quella di non minimizzare i cambiamenti climatici degli ultimi anni, diffidando però delle previsioni catastrofiche. Senz'altro occorre portare avanti le buone pratiche per inquinare meno, risparmiare energia e potenziare le fonti rinnovabili, e questo a prescindere dagli effetti dei gas serra. Le politiche ambientali sono legate da una parte al sistema di informazione, educazione e sensibilizzazione del cittadino verso le tematiche ambientali e, dall'altra, al controllo delle emissioni, con particolare riferimento all'abbassamento delle emissioni degli inquinanti atmosferici generati dagli impianti industriali, dai mezzi di trasporto e dagli impianti termici ed energetici. A sostegno di una crescita economica galoppante dagli inizi degli anni '90 che vede aumenti superiori del 20 per cento dei consumi mondiali del petrolio e aumenti superiori al 60 entro il 2030 della domanda di energia, occorrono azioni dirette a garantire la sostenibilità futura, in particolare in ordine al contenimento delle emissioni dei gas serra, al miglioramento della qualità dell'aria (specialmente nelle aree urbanizzate e nelle aree naturali protette), alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla sicurezza energetica, con particolare riferimento alla diminuzione della dipendenza dell'Italia dalle importazioni. Ma per raggiungere tali obiettivi non servono accordi burocratici, aprioristici e unilaterali; ciò implica la necessità di una politica di rinnovo delle fonti energetiche del Paese diretta alla transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi energetici sostenibili. Si tratta di valutare soluzioni intelligenti che siano soddisfacenti per la lotta ai cambiamenti climatici ma anche per la sicurezza energetica e l'occupazione che non penalizzino il nostro Paese in termini economici. Nell'ambito di tali sistemi deve trovare assolutamente spazio, ad esempio, l'utilizzo dell'idrogeno per la produzione di energia elettrica su vasta scala e, senz'altro, la rivalutazione dell'energia nucleare, anche al fine di non escludere l'Italia dagli scenari futuri degli investimenti europei in questi settori. L'Accordo europeo dell'anno scorso sul 20-20-20 (che 20-20-20 (che comporta una riduzione dei gas ad effetto serra del 20 per cento rispetto al 1990, una riduzione dei consumi energetici del 20 per cento, attraverso un aumento dell'efficienza energetica e l'uso dei biocarburanti per il 10 per cento della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti, e l'ampliamento della quota di energie rinnovabili sul consumo energetico finale dell'Unione europea del 20 dell'Unione europea del 20 per cento) è estremamente penalizzante per l'economia del Paese e per lo sviluppo delle nostre imprese. Proprio per questo è stata chiesta ed ottenuta in sede di Unione europea una revisione degli accordi nei

il Governo deve promuovere a livello europeo una revisione degli accordi già stipulati, che possano rivedere le politiche ambientali, energetiche ed industriali dell'Unione europea. Lo sviluppo delle potenzialità del sistema europeo verso un'economia verde e decarbonizzata deve basarsi piuttosto sulla revisione degli standard di efficienza energetica, soprattutto con riferimento alle fonti rinnovabili e al nucleare, sulla ridefinizione della fiscalità energetica, sull'istituzione di misure armonizzate per la valorizzazione di settori come quello agro-zootecnico o quello della gestione delle foreste. I nuovi accordi devono contenere misure fiscali e finanziarie di supporto alle imprese; anzi, l'obiettivo principale deve essere quello di evitare penalizzazioni per le imprese e gli investitori nel mercato europeo ed internazionale, allo scopo di incentivare

che impegna il Governo nella direzione di una revisione degli accordi europei già stipulati. Signora Presidente, ho chiesto di intervenire in questo dibattito che considero molto rilevante, per fare qualche considerazione di carattere politico.

Rilevo che sono passati pochi giorni dal momento in cui il Presidente del Consiglio - mi sembra l'abbia ricordato anche il presidente D'Alì - ha fatto vanto di essere riuscito a imporre con la sua forza politica al nostro Paese una visione, com'è stato detto, negazionista del problema. Si è fatto vanto di avere imposto al Paese una visione secondo la quale i problemi climatici non esistono: i problemi dell'inquinamento, del cambiamento del mondo

su quali basi scientifiche questa posizione si fondi. Questa mattina nella discussione delle mozioni sulla corruzione ho sentito esprimere la tesi - per me, scusatemi, stupefacente - che alla corruzione non ci si oppone

possa permettersi di contrastare la corruzione senza controlli e senza sanzioni, sottolineo, adeguati.

al problema del clima noi rispondiamo coltivando la libertà. Pochi giorni fa un

una campagna su come possa essere l'Italia nel 2050. Ha esordito parlando dei temi di casa sua; si tratta di un giornale di proprietà della Confindustria, quindi ha proposto le questioni che stanno a cuore all'Italia produttiva: meno burocrazia, infrastrutture, ricerca e fondi per la ricerca, un fisco meno *killer*, un federalismo fiscale reale e non sloganistico, un piano energetico di nuova generazione. Riotta non ha citato nel suo editoriale, in vista del 2050, i problemi ambientali. Ecco, io credo che se noi smettessimo di pensare soltanto a quello che succederà nelle prossime ore e ci dessimo una visione più ampia e pensassimo al futuro del nostro Paese,

preparazione del nostro Paese al futuro avrebbe una posizione prioritaria nella nostra attività politica. Voglio dirlo in modo chiaro: io non ho la competenza per trattare il problema in termini scientifici, ma vorrei sottolineare le questioni politiche che mi sembrano più rilevanti rivolgendomi ad un interlocutore della maggioranza di cui conosco la sensibilità su alcuni aspetti della vita del nostro Paese. Considera mai la Lega Nord quali saranno gli effetti

Si rende conto la Lega Nord di quale sarà la massa di immigrazioni che si riverserà in Europa e prima di tutto in Italia? Si rende conto che non prendere misure adeguate per la difesa del clima e per contrastare una tendenza che appare irreversibile è un delitto proprio per chi pone come problema prioritario la vastità del fenomeno immigratorio? Si rende conto la Lega Nord che la migliore prevenzione di quello che è stato il primo problema su cui ha costruito le proprie fortune politiche è proprio una buona politica in materia di clima?

se aveste potuto risparmiare le risorse che avete dovuto impiegare per rimediare ai problemi provocati dal clima. Per non parlare della salute: io mi dolgo di non vedere qui presente il Ministro dell'ambiente perché penso che quando un ramo del Parlamento, il Senato in particolare, discute di materie climatiche il Ministro dell'ambiente dovrebbe essere in Aula, ma devo dire anche che mi dolgo di non vedere il Ministro della salute perché anch'egli dovrebbe essere presente in Aula quando si dibattono problemi di questo genere. Signora Presidente,

onorevoli colleghi, anche noi consideriamo estremamente importante la materia che stiamo trattando questa mattina.

criticare, ridicolizzare le mozioni degli altri, e soprattutto la nostra. Siamo un po' abituati a questo approccio spocchioso e supponente da parte vostra; personalmente cerco di intervenire spiegando qual è il nostro punto di vista e chiedendo rispetto. Vedete, noi non siamo negazionisti. Non mi riconosco in quel termine, che peraltro mi fa venire in mente situazioni e valutazioni completamente diverse e agghiaccianti. Noi siamo per conoscere meglio le questioni sulle quali dobbiamo decidere, per non piegarci ad un'opinione pubblica mondiale pesantemente manipolata. Abbiamo, o cerchiamo di avere, un approccio antidogmatico e non ideologico, sostanzialmente laico. come ridicoli agli occhi del mondo. Meno male - mi è venuto da pensare mentre ascoltavo questo mio collega - che c'è la sinistra in Italia che ci difende da questa lettura ridicola della politica del nostro Paese, quando si impegna per evitare il nucleare, quando si impegna per evitare la realizzazione dei treni ad alta velocità, quando si impegna per evitare la realizzazione degli inceneritori (quindi ci espone al ridicolo nel mondo, quello sì).

e molta confusione, non solo sui media, ma anche nelle aule parlamentari. Anche negli autorevoli interventi di questa mattina troppi colleghi hanno confuso la complessità dell'argomento climatico con la complessità degli argomenti di politica ambientale. Politica ambientale non vuol dire solo politica sul clima. La politica ambientale è molto più ampia: dentro c'è anche il clima; pure, inquinamento non vuol dire CO2. Abbiamo, infatti, diffuso - questa mattina lo abbiamo ripetuto più volte ed è anche scritto, e questo è particolarmente preoccupante

perché qualcuno magari le legga. La CO2 non è un inquinante. La comunicazione - e ahimè anche la politica - confonde spesso le emissioni di CO2, che potrebbero avere influenza sulle dinamiche del clima, con le emissioni inquinanti, che hanno certamente effetti nefasti sulla salute degli uomini, degli animali e delle piante. Questi vanno combattuti. Noi non siamo contro le politiche ambientali: siamo contro la politica ambientale che drena risorse che sarebbero indispensabili contro l'inquinamento chimico-fisico correre dietro a un'ipotesi (che oggi è ancora un'ipotesi) di incidenza delle emissioni antropogeniche di CO2 sulle dinamiche complesse del clima, che non conosciamo ancora a fondo. Quindi noi non siamo contro le politiche ambientali: siamo per una diversa politica ambientale. Grazie alla CO2, dicevo prima, le piante svolgono la fotosintesi (pensate un po', lo abbiamo imparato a scuola), reazione in virtù della quale sei molecole di CO2 e sei molecole di acqua producono una molecola di glucosio (zucchero) e una molecola di ossigeno. Questa semplice reazione avviene sfruttando l'energia solare ed è alla base della vita sul nostro pianeta. Può essere banale dirlo, ma va ripetuto, perché altrimenti i nostri cittadini pensano che la CO2 sia un mostro chimico che ci sta uccidendo. È un'altra cosa: i mostri chimici che ci stanno uccidendo continuano ad essere emessi, sversati nei mari e negli oceani e sono in circolo su tutto il pianeta. Un altro difetto è quello della semplificazione. Il clima - vedete, colleghi - non è semplicemente rappresentabile con la temperatura, e non è mai stato stabile. Per sua natura è mutevole, ed è uno dei motori dell'evoluzione del pianeta. Abbiamo prove geologiche sulla sua variabilità passata, talmente numerose che davvero sembra impossibile ignorarle. Senza andare alla geologia, per rispondere al catastrofismo del collega Zanda e ai danni da lui evocati, credo che girando in qualsiasi nostro borgo troviamo delle targhe del 1700 o del 1800 dove viene indicato il livello magari di quel corso d'acqua, di quel rio, di quel torrente che allora esondò facendo morti e danni. Quindi, non diciamo ai nostri cittadini che per il clima in passato vi era una sorta di età dell'oro, che vi era una sorta di «mondo del Mulino Bianco», dove il clima non faceva danni, dove la natura non aveva i suoi corsi e i suoi ritmi e non creava problemi problemi alle comunità umane. Non spieghiamo questa verità che non esiste; spieghiamo che la natura è da sempre un pericolo, che non è l'uomo che l'ha destrutturata e l'ha modificata, ma è l'uomo che deve avere il senso di responsabilità di governarla. il clima è qualcosa di molto più complesso, comprende molte variabili, quali ad esempio l'umidità atmosferica, la radiazione solare, in tutte le sue componenti e la circolazione atmosferica che lega tutti questi aspetti. Troppe ricerche restringono lo studio del clima ad una sola variabile, la temperatura. In ogni caso, anche l'effetto serra è considerato indispensabile per garantire

un effetto serra che non esagera, non esorbita nelle sue funzioni è indispensabile per la vita nel pianeta. Come dicevo, il clima è determinato in gran parte dal vapore acqueo e dalle nubi, come spiegava bene in precedenza il presidente Possa. Insieme sono responsabili dell'80 per cento

capite - ma cercherò di illustrarlo successivamente - come sia ininfluente lo sforzo che ci stiamo impegnando a fare a livello europeo. Riteniamo quindi che sia indispensabile continuare, anzi aumentare gli sforzi nella ricerca scientifica per capire il sistema climatico: è indispensabile per la vita dell'uomo sul pianeta. Quindi, continuiamo ad investire in ricerca, aumentiamo questa nostra capacità di comprendere i meccanismi complessi delle dinamiche climatiche. (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) non è una ONG (questo è un piccolo divertimento). Assistiamo - e mi fa sorridere - ad una sinistra che da sempre in qualche modo critica gli organismi governativi ed enfatizza le ONG. Qui abbiamo un organismo intergovernativo che viene glorificato dal centrosinistra; è l'eccezione che fa la regola.

fondamentali, sono le Tavole della Bibbia. Capite quindi come il nostro approccio provinciale rispetto a questi termini, a queste sigle, che tanto riempiono la bocca ai nostri colleghi di centrosinistra, ci fa sorridere, perché io credo che il nostro Parlamento abbia il dovere di esprimere un punto di vista, anche se quest'ultimo alle volte può essere un po' dissonante con quello che i Governi mondiali discutono a livello centrale. Insomma, colleghi, spesso veniamo rimproverati di essere succubi dell'azione di governo, di essere un votificio. A me pare invece che quelle poche o tante volte nelle quali ci permettiamo di esprimere un nostro punto di vista, e lo facciamo con garbo, lo facciamo cercando di spiegare le nostre ragioni, siamo luogo ridicolizzati perché non ci adeguiamo a questo modo globale e appiattito sulle posizioni dell'IPCC di accettare queste dinamiche e queste politiche; in secondo luogo siamo criticati perché abbiamo osato dire qualcosa un po' dissonante rispetto alle scelte fatte dal Governo. Ma voi dovreste applaudire questa nostra posizione perché oggi, come altre volte, dimostriamo una nostra autonomia! Chiediamo in qualche modo al nostro Governo di ascoltarci; chiediamo anche noi al Ministro dell'ambiente di venire in Aula ad ascoltare questo dibattito. Ci farebbe piacere approfondire con il nostro Ministro, prima che vengano assunti accordi a livello internazionale, argomenti importanti per il nostro futuro, come questo. Mi pare di ricordare - ma potrei sbagliarmi - che queste posizioni non sono scritte nel programma di governo del centrodestra che è stato votato dagli italiani; c'era il nucleare, certo che sì, ma tutte queste scelte sulla lotta al *global warming*, tutte queste scelte che ci chiedono di indirizzare risorse importanti per il nostro sviluppo in questo momento su queste tecnologie, e magari non su altre, io non le ricordo nel nostro programma. Sarebbe allora buona cosa che, grazie anche allo stimolo che cerchiamo di dare questa mattina, si potesse aprire un ulteriore confronto, ancora più approfondito, su questi argomenti. l'Unione europea, e in particolare l'Italia, proprio basandosi su queste posizioni discutibili del'IPCC che hanno dimostrato, anche attraverso il cosiddetto scandalo climagate, di non essere così affidabili, ha assunto posizioni e politiche unilaterali rispetto al resto del mondo molto impegnative e costose. La mancata assunzione di impegni vincolanti al vertice di Copenaghen da parte dei Paesi maggiori produttori di CO2, la Cina in testa, come hanno detto molti colleghi che mi hanno preceduto, e la sempre e la sempre maggiore perplessità sull'affidabilità delle analisi dell'IPCC rendono inutili queste misure in termini di incidenza sul sistema clima. Quindi, spenderemmo molto danneggiando molto le nostre economie per incidere sostanzialmente quasi nulla, perché scarsa è la nostra incidenza sulla produzione mondiale di CO2 e scarsa è la nostra conoscenza delle dinamiche del clima. Fatte queste premesse, come è stato illustrato prima, invitiamo semplicemente il nostro Governo a valutare la possibilità di chiedere in sede ONU di rivedere gli assetti degli organi che hanno determinato queste strategie sbagliate, di riorganizzare l'IPCC (facendo sì che sia maggiormente un organo scientifico

di valutare la possibilità di chiedere la sospensione di progetti dell'Unione europea che risultino particolarmente onerosi per le casse europee e basati su queste errate previsioni dell'IPCC. Lo ripeto, le politiche ambientali non sono esclusivamente le politiche climatiche, e noi non ci stiamo a farci schiacciare nel ruolo dei negazionisti e di quelli che non hanno a cuore il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti e dell'ambiente nel quale viviamo. Non siamo d'accordo a spendere troppe risorse pubbliche su un argomento come quello dei mutamenti climatici che non è chiaro, drenandole invece dalla lotta dell'inquinamento chimico-fisico che è chiaro e che produce milioni di morti all'anno.

seguo l'ordine che mi è stato indicato e, data la complessità della materia, mi esprimerò per ogni mozione, sui singoli punti del dispositivo. Inizio dalla mozione n.

una premessa. Noi abbiamo una visione realistica dei cambiamenti climatici, non vogliamo aderire alle posizioni dei catastrofisti che utilizzano la paura per portarci su certe strade, ma non siamo d'accordo con coloro che fanno finta di niente; i qualunquisti rischiano di indurci a non affrontare i problemi. Siamo indubbiamente consapevoli che il problema debba essere affrontato conciliando la tutela dell'ambiente con lo sviluppo e, sebbene su alcuni punti la nostra posizione sia differente da quella della maggioranza, specie per quanto riguarda il cosiddetto Accordo 20-20-20, pensiamo sia importante ed apprezzabile l'impegno che si sta assumendo in materia di cambiamenti climatici. In particolare, la mozione presentata dai colleghi del Popolo della Libertà sottolinea la necessità di adoperarsi affinché la politica dell'Unione europea si incentri su emergenze planetarie concretamente affrontabili e nell'elaborazione di progetti che contengano certezze sul rapporto costi-benefìci. Pensiamo che questo sia un atteggiamento realistico, ragionevole e sostanzialmente lo condividiamo. Allo stesso tempo, siamo d'accordo con i colleghi dell'Alleanza

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, l'accordo raggiunto a Copenaghen, pur in assenza dell'auspicata nuova intesa vincolante sulla riduzione di gas serra, parte dal definitivo riconoscimento del fatto che i cambiamenti climatici sono una delle più grandi sfide del nostro tempo, sottolineando l'urgenza di un intervento su questo fronte ed introducendo a tal fine, per la prima volta formalmente, l'obiettivo di evitare il superamento dell'aumento di due gradi delle temperature del pianeta. Si tratta di un accordo internazionale che il Governo italiano ha sottoscritto e che quindi deve onorare, anche perché richiama espressamente l'articolo 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, di cui il nostro Paese è parte. I trattati internazionali si onorano. I patti si rispettano. Gli accordi si mantengono. Ovviamente, questo non significa che si debba rinunciare a migliorarli agendo nelle sedi opportune. Ci si può dividere sul punto di vista di ciò che consiste in un miglioramento, ma non si può ignorare, come fa la mozione n. 248 del senatore D'Alì, che l'Italia ha aderito agli obiettivi di riduzione volontari comunicati dall'Unione europea il 31 gennaio scorso. Pochi giorni fa il Segretariato della Convenzione quadro dell'ONU ha pubblicato il rapporto ufficiale sui risultati della Conferenza di Copenaghen del dicembre 2009, dal quale emerge che 75 Paesi aderenti alla Convenzione hanno trasmesso i loro obiettivi nazionali sulla riduzione delle emissioni entro il 2020. Il rapporto contiene il testo dell'Accordo di Copenaghen e la lista delle 112 parti (111 Stati più l'Unione europea) Come si vede, mancano ancora oltre 80 firmatari, ma risulta evidente che la comunità internazionale ha da tempo concordato sulla gravità del problema e sui rimedi necessari a farvi fronte.

non possiamo disinvoltamente negarla, se non sconfessando anche la scienza e i Governi italiani - tutti i Governi - che questa certezza hanno saggiamente preso in considerazione. Non si tratta quindi di dividersi secondo vecchie linee ideologiche preconcette che l'Accordo di Copenaghen, con tutti i suoi limiti, ha definitivamente superato. Con diversi accenti, anche in Italia tutti i Governi hanno, almeno a parole, riconosciuto l'importanza di proseguire nella concreta partecipazione e nel fattivo sostegno alla formazione ed attuazione delle iniziative europee volte al controllo e alla riduzione delle emissioni inquinanti. Si può dissentire sui costi, sui tempi, sui meccanismi, ma non sull'essenza stessa del problema, a meno di non voler gettare l'Italia in un isolamento che, oltre ad essere politicamente incomprensibile, sarebbe economicamente deleterio. Tutti i Governi si sono detti disposti a proseguire nell'adozione di misure a sostegno degli investimenti all'innovazione, alla ricerca ed allo sviluppo delle tecnologie pulite,

Tutti i Governi e le parti politiche possono concordare con l'obiettivo di promuovere ulteriormente, con particolare riferimento al settore edilizio e a quello dei trasporti, gli interventi diretti al risparmio energetico e all'efficienza energetica, compresa l'efficienza delle reti. Riteniamo, quindi, necessario un impegno del Governo a procedere nelle politiche ambientali e di contrasto al cambiamento climatico, assicurando anche il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle politiche di ricerca e sviluppo,

poiché si situano in un alveo internazionale consolidato, sia sul piano delle buone pratiche concrete cui anche il Governo italiano si deve richiamare. Dopo Copenaghen resta l'obiettivo definito nella cosiddetta *Road map* di Bali, così come restano aperti e da definire ulteriori nodi negoziali che dovranno essere discussi e deliberati nei prossimi mesi. Il Consiglio europeo ha affrontato, tra le altre cose, la questione dell'avanzamento dei negoziati per un accordo globale sui cambiamenti climatici ed i Capi di Stato e di Governo hanno convenuto sull'esigenza di una nuova dinamica nel processo negoziale della Convenzione. L'Unione europea si è dichiarata pronta a fare la sua parte mantenendo gli impegni presi a Copenaghen, proprio in vista delle prossime sessioni di Bonn e Cancun. La consapevolezza dell'importanza del tema per le pubbliche opinioni di tutto il mondo è una rilevante eredità di Copenaghen. Particolarmente forte l'impegno assunto dai Paesi in via di sviluppo per le rinnovabili. L'accordo ha il pregio di costringere i Paesi ad indicare i propri impegni, che potranno essere rivisti, confermati o migliorati nel corso del 2010. Il rispetto della scadenza del 31 gennaio non ha avuto unicamente una valenza formale, ma ha significato che il processo negoziale è destinato a continuare durante tutto il 2010. Ben 119 su 192 Paesi, in rappresentanza di oltre l'80 per cento delle emissioni globali, hanno comunicato volontariamente i loro impegni. Nelle conclusioni approvate a fine marzo dal Consiglio europeo si legge che tra «gli obiettivi comuni che guidano l'azione degli Stati membri» per la strategia economica Europa 2020 c'è anche quello di «ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990», aumentando al contempo al 20 per cento la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico finale e puntando ad un miglioramento del 20 per cento dell'efficienza energetica, così come stabilito dal vigente pacchetto clima-energia. L'obiettivo supplementare dell'Unione europea è quello di ridurre le emissioni del 30 per cento entro il 2020, a condizione che gli altri Paesi industrializzati facciano sforzi comparabili. L'Unione europea ha dunque confermato il proprio obiettivo di riduzione delle emissioni del 20 per cento al 2020 e condiziona un ulteriore taglio del 10 per cento ad un accordo globale, ma il dato rilevante è l'alta percentuale di emissioni che i Paesi impegnati rappresentano. Anche se un gruppo limitato di Paesi, che tuttavia rappresenta un'elevata percentuale delle emissioni globali, riesce a negoziare un accordo efficace, l'obiettivo si può dire in buona parte raggiunto. Il negoziato sui cambiamenti climatici non può essere fermato, poiché resta estremamente complesso. Non vi è solo infatti la riduzione delle emissioni attraverso le politiche di mitigazione, ma anche il tema della deforestazione, dell'uso del suolo, la questione dei finanziamenti aggiuntivi alle azioni di adattamento delle regioni più povere e vulnerabili. C'è infine la questione della verifica e dell'osservanza degli impegni. Concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei valori sulla mozione n. 260 e su quelle mozioni che intendono promuovere le azioni internazionali sul clima e sulle energie rinnovabili, nel rispetto degli impegni assunti e degli accordi internazionali.

Il Senato sta diventando, per iniziativa certamente rimarchevole di alcuni colleghi del PdL, un luogo in cui si svolge a scadenza periodica un dibattito di natura scientifica. Non so se sia proprio compito del Senato fare dibattiti di natura scientifica per

per non metterla completamente in rotta di collisione con le posizioni che il Governo Berlusconi assume a livello internazionale.

ed è significativo che nessuno, neanche tra i collaboratori del Governo, se ne sia accorto - la mozione che abbiamo presentato riprende letteralmente e testualmente un certo documento politico. Mi al documento che così inizia: «Noi leader del G8, incontrandoci all'Aquila, esprimiamo la nostra solidarietà dal più profondo del cuore al popolo dell'Abruzzo, colpito dal tragico terremoto che ha investito la regione il 6 aprile 2009 e a tutti coloro che nel mondo sono stati toccati da disastri naturali».

ripeto - dal Governo italiano e sottoscritti dal Governo Obama e da tutti i Governi che hanno partecipato al G8 dell'Aquila. Questo documento contiene alcuni paragrafi concernenti i temi del clima e dell'ambiente. Essi sono la nostra mozione. Quindi, la sottosegretario Ravetto ha espresso un parere critico su un testo che è letteralmente quello presentato dal Governo Berlusconi e dai leader riuniti all'Aquila nell'occasione che, comprensibilmente e anche giustamente, il Governo reputa come una delle sue più prestigiose riuscite. Oggi l'Aula del Senato, venisse confermata questa impostazione, si troverebbe a bocciare il documento che il Presidente del Consiglio ha presentato all'Aquila ed ha approvato e che, per così dire, è stampato e distribuito.

sono emersi alcuni elementi critici e, soprattutto, è emersa da parte di quel gruppo qualificatissimo di ricercatori - il migliore al mondo - una preoccupazione al confronto scientifico e alla trasparenza del dibattito scientifico che è affiorata nella celebre vicenda che alcuni colleghi hanno rievocato

dei documenti prodotti da quella comunità scientifica a una loro radicale bocciatura, in totale contrasto con quello che poi da domani il Governo italiano sarà chiamato a dire nelle sedi internazionali, è non solo sbagliata, ma, come ben si può comprendere, del tutto contraddittoria. Mi permetto di dire alla sottosegretario Ravetto che i tre punti sui quali ha espresso parere contrario contrario sono letteralmente tratti dagli impegni scritti dal Governo Berlusconi all'Aquila in occasione del G8 a guida italiana, a guida del Governo di cui lei fa parte.

come strumento per accelerare l'integrazione efficiente e sicura delle fonti di energia rinnovabile e della generazione distribuita nel sistema elettrico e per migliorare l'efficienza energetica; a sostenere i lavori attualmente il paragrafo 88, lettera *c)*, del documento dell'Aquila, dove addirittura il nostro Governo premette che si impegna -

È quella approvata nelle mozioni della Camera dei deputati, che hanno un segno completamente diverso? O è quella che cercate di far passare ostinatamente al Senato? Non è meglio, sottosegretario Ravetto, trovare una definizione ragionevole di compromesso? Tenete conto che su queste materie vi ritroverete da domani a dover operare facendo parte dell'Unione europea - perché fino a prova del contrario continuerete e continueremo a farne parte - e di una comunità internazionale che si riconosce in documenti come quelli che sono tradotti nella nostra mozione per mettervi alla prova. Potete respingere

mi auguro che il Governo ci ripensi velocemente, e non solo si rimetta all'Assemblea, ma dia anche un parere favorevole rispetto alle posizioni che esso stesso ha assunto a livello internazionale. *(Applausi Grazie, Presidente, la Lega Nord ha da sempre sostenuto tutte le misure prese dal Governo: quelle verso la promozione dei legittimi interessi nazionali nel negoziato in sede europea e internazionale per la lotta ai mutamenti climatici, salvaguardando gli interessi delle imprese italiane ed evitando penalizzazioni; verso il sostegno della ricerca per l'innovazione tecnologica ed il risparmio energetico; quelle verso le politiche innovative nel settore dei trasporti e della mobilità, anche per abbattere l'inquinamento da polveri sottili che particolarmente affligge i nostri territori padani; verso le incentivazioni per la sostenibilità energetico-ambientale dei programmi edilizi. Chiaramente, però, non possiamo accettare i discorsi catastrofisti mossi dall'eccessiva percezione dello spettro del riscaldamento globale, che hanno portato ai vincoli aprioristici dell'Accordo del 20-20-20, impegni che inevitabilmente finiranno per penalizzare le nostre imprese, specialmente in questo momento di drastico deterioramento degli scenari macroeconomici internazionali. Le più recenti valutazioni degli esperti sulla situazione mondiale del clima hanno dimostrato che gli annunci catastrofici di qualche mese fa non sono confermati da dati scientifici. E se le analisi effettuate fino ad oggi si sono rivelate errate è evidente che occorre un cambiamento sostanziale della politica di intervento; in altre parole, occorre ripensare le strategie per la mitigazione del rischio da riscaldamento globale. Lo Stato, ma anche l'Europa, ha l'obbligo di trovare un punto di equilibrio, conciliando l'esigenza di promuovere i sistemi produttivi, ovviamente in termini compatibili con la tutela dell'ambiente, ma anche con la strategia di non imporre agli stessi sistemi produttivi oneri oneri eccessivamente gravosi. Secondo noi il Governo deve promuovere a livello europeo una revisione degli accordi già stipulati, così da rivedere le politiche ambientali, energetiche ed industriali dell'Unione europea. I nuovi accordi devono contenere misure fiscali e finanziarie di supporto alle imprese. Anzi, l'obiettivo principale deve essere quello di evitare penalizzazioni per le imprese e per gli investitori nel mercato europeo e internazionale, allo scopo di incentivare e rinforzare le forze economiche e irrobustire l'economia reale. Occorre porre fine alla nuova burocrazia internazionale che si sta creando in tema di cambiamenti climatici. L'Europa dovrebbe dedicarsi piuttosto alla promozione di progetti internazionali per affrontare la sfida tecnologica globale valorizzando tutte le potenzialità della nostra economia integrata, che ha già raggiunto livelli significativi di efficienza e innovazione. Occorre costruire una nuova economia globale in grado di sostenere la crescita e ridurre le emissioni attraverso i suoi punti di forza che sono quelli dell'efficienza energetica, della promozione delle fonti energetiche rinnovabili e del nucleare, ma anche della migliore gestione delle foreste, accompagnati da proposte concrete sulle misure finanziarie e sulle regole internazionali necessarie per sostenerle. Tali azioni devono essere fortemente incentrate su politiche volte ad accelerare l'innovazione e la diffusione tempestiva di nuove tecnologie e infrastrutture che permettano così di creare un margine competitivo per le imprese italiane nei settori chiave del futuro: mi riferisco soprattutto ai settori dell'efficienza energetica, automobili verdi, reti intelligenti, tecnologie per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica, energie rinnovabili, conservazione e promozione degli ecosistemi. Nel complesso, il nostro Gruppo ritiene che occorra una revisione profonda delle politiche europee sulle politiche ambientali, che deve iniziare proprio dalla revisione del cosiddetto Accordo del 20-20-20 sui cambiamenti climatici, e ritiene opportuno un impegno del Governo in tal senso. Pertanto, il Gruppo

nove clandestini, migranti ghanesi e nigeriani, sono stati praticamente sequestrati per giorni e notti in una nave

chiedendo alla nave di ripartire verso Genova, dove probabilmente sarebbero stati nuovamente cacciati via e quindi riportati in Costa d'Avorio, dove non potevano neanche essere accolti perché sprovvisti di documenti.

Nel frattempo che questa richiesta viene valutata ed esaminata dalle autorità competenti, è stato emesso contro di loro un decreto di respingimento, il quale, come recita la legge più attuale su tale questione, deve essere sospeso in attesa della valutazione sulla richiesta di asilo. mio Gruppo, che sia prevista e rispettata la procedura della legge, senza un intendimento persecutorio verso queste persone,